L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847,

Non si tratta di soglie qualsiasi.

non superiore al 4 per cento dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica». Ciò vuol dire avere quel minimo di scostamento tra valutazioni che possono essere effettuate da un determinato tecnico (tutti sapete che le valutazioni possono oscillare dagli uni agli altri) e avere qui una determinazione precisa di quella che è l'alterazione del risultato economico di esercizio tale da determinare la certezza. Signor Presidente, lei mi insegna che se un'impresa straniera

L'avvocato cosa risponde? Stando alle parole del relatore, dipenderà dall'interpretazione della giurisprudenza. Quanto al nostro compito, si è detto ieri che non compete a noi dare interpretazione. No! A noi compete dare certezza alla norma penale, alla condotta, all'evento, al dolo e a tutti gli elementi della fattispecie. La certezza è tale da incidere sul problema della vita delle aziende e sul problema della vita degli degli investimenti che le società vogliono fare in Italia. Quindi, ci troviamo davanti ad una fattispecie che viene integrata *ad libitum* da qualsiasi giudice. Ognuno farà le proprie valutazioni sulla rilevanza o meno. Aspetteremo anni - lei mi insegna - per avere una giurisprudenza sedimentata o un pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione che ci diranno cosa vuol dire Mi si deve dunque spiegare perché non individuare dei livelli chiari e precisi di non punibilità. Le soglie attualmente vigenti sono state ritenute conformi e legittime dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte costituzionale italiana. Anzi, la nostra Corte costituzionale ha detto una cosa chiara e sacrosanta: servono a delimitare il potere di interpretazione dei giudici e a dare contezza e certezza del precetto normativo, che devono essere mantenute. Non intendo mantenere le soglie attualmente vigenti

invece ragionando sulla certezza del precetto penale e abbiamo ragionato su tutta questa normativa. Ha visto che

proprio ieri, in un convegno, ha messo in evidenza come la corruzione sia un problema che va combattuto, specialmente attraverso la prevenzione.

di definizione della fattispecie penale, si propone quindi di tornare a delle soglie, che non sono quelle attualmente vigenti, ma che hanno la possibilità di essere valutate concretamente, determinando finalmente una certezza. se dobbiamo approvare una norma che non avrà efficacia immediata, perché dobbiamo attendere l'interpretazione della giurisprudenza al fine di dare la valutazione dell'esatta portata,

se una spiegazione non c'è, vuol dire che avete fatto una norma manifesto, ovvero che volete soltanto sbandierare una norma senza raggiungere alcun risultato.

con quei commi che i miei emendamenti si propongono di abrogare, si mette in atto un prolungamento, ingiustificato dal punto di vista della normativa comunitaria e delle norme sulla concorrenza,

la corruzione va combattuta: in questo quadro è necessario cancellare o modificare le norme che consentono, addirittura magari a norma di legge, di fare proprio quello che con questo provvedimento stiamo cercando di evitare, e cioè che ci siano guadagni o profitti da parte di qualcuno in un regime di disparità. Allora, se un'azienda, piuttosto che un privato, acquisiscono dei lavori dallo Stato, dal Comune o da una pubblica amministrazione

invitare l'Aula a dare un'interpretazione alla norma. Ieri, infatti, il relatore ha detto che non compete al Senato stabilire se le «valutazioni» fanno o meno parte dei fatti non rispondenti al vero.

Noi non possiamo rimettere il giudizio alla giurisprudenza perché, se diciamo questo, veniamo meno al nostro compito: il giudice,

Vi rendete conto delle abnormità commesse nel corso dei lavori di questo Senato? Signor Presidente, io credo che lei abbia il dovere di chiedere ai Gruppi di esprimere la propria opinione.

per la dignità di questa Aula e del Parlamento e per lo svolgimento del lavoro che gli compete, cioè dare norme chiare e precise. Non possiamo delegare ad altri addirittura che la norma diventi incostituzionale, secondo quanto la stessa Corte costituzionale ci ha sempre insegnato. Non può essere il giudice a delimitare la fattispecie penale. Nell'ipotesi di specie voglio sapere da ciascun Gruppo, che si assume così la propria responsabilità politica, se ritiene di rimettere al giudice l'interpretazione: le valutazioni rientrano o non rientrano?

non vorrei far cadere nel nulla l'appello del collega Caliendo, perché va al nocciolo della questione politica: o vogliamo fare il nostro mestiere o lo deleghiamo sostanzialmente ad altri.

Si parla di dignità della persona che non può essere tenuta in un processo all'infinito, *sine die*? Allora tutto il sistema parlamentare

o, comunque, minimali rispetto alla struttura societaria, al bilancio della società possono essere - per così dire - perdonati, sanati,

stabilita con norma. Il Governo stabilisce questo principio, ma poi qualcuno avverte il *Premier* che andrebbe a definire, a chiudere alcuni processi a carico del suo massimo esponente nonché avversario politico.

stiamo facendo il lavoro di legislatori nel peggiore dei modi. *(Applausi

efficaci. Il Governo ha deliberatamente cancellato e messo la scolorina - è un Governo che, con le scolorine, ci sa fare - sulla locuzione «ancorché oggetto di valutazioni».

costruito unicamente su valutazioni: la valutazione dei crediti di una banca, l'incaglio, la sofferenza, l'esigibilità, la valutazione del valore di un immobile. il Governo e il relatore ci vogliono spiegare in che modo intendono verificare la mancanza di questa formulazione, che era ben espressa nella locuzione previgente degli articoli del codice civile che ho testé elencato e che sono - lo ripeto - il 2621, il 2622 e il 2638? Hanno una spiegazione logica plausibile

sia del relatore che del Governo, perché questo emendamento tende semplicemente a rendere coerente la formulazione. Nel testo si fa riferimento alle «falsità», mentre in altri provvedimenti di legge si definisce il comportamento in questione

Signor Presidente, non riesco a capire le motivazioni del parere contrario espresso su questo emendamento. Se noi prevediamo il falso in bilancio per le società quotate e non quotate, non capisco perché non possiamo prevederlo per le fondazioni.

Qualche settimana fa, il Presidente di Confindustria ha messo in guardia contro i pericoli insiti in alcune parti del provvedimento

mettere le aziende in mano non solo ai singoli magistrati, i quali singolarmente possono prendere dei provvedimenti che, anche se poi non confermati in sede di giudizio,

al di sotto del quale non si incorre in tali reati, opinabilmente diverse, perché sappiamo che in tutti i campi ci sono questioni che sono materia di opinione tra i vari esperti, anche nella massima buona fede, e naturalmente ciò avviene anche in sede di bilancio.

a pene molto pesanti, e non per un attivo tentativo di creare imbrogli, di commettere reati, di danneggiare soci o di sottrarre quanto dovuto al fisco,

L'emendamento proposto dal senatore Galimberti - peraltro uomo del settore dell'imprenditoria e del commercio e, quindi se questo è l'unico emendamento che ha presentato, ci sarà pure una ragione

ha a che fare con la pubblica amministrazione. Se si cerca l'appesantimento delle pene e l'aumento della minaccia dal punto di vista quantitativo,

proviamo a dire che non c'è un intento punitivo o la volontà di far scappare all'estero le aziende. C'è la volontà di far rispettare le norme, che prevedono anche di fare un bilancio corretto, ma non di

che era fiore all'occhiello nel mondo e ci sarebbe stata una fuga verso posti barca all'estero e molti

situazione si aggraverà perché sta già succedendo. Non c'è una delocalizzazione nei Paesi dell'Est o del Nord Africa, ma nelle avanzate Nazioni come la Svizzera, l'Austria e la Francia. il mettere un limite non superiore al 10 per cento, che il relatore e il Governo potrebbero anche riformulare e ridurre, significa impedire che si verifichi proprio la fuga delle nostre imprese, con conseguente aumento della disoccupazione. Noi ve lo abbiamo detto e poi ve lo rifaremo rivedere, come é successo per la nautica. Prima o poi il popolo italiano capirà chi ha ragione o torto, chi fa l'interesse del suolo, dell'occupazione e dello sviluppo chi invece ne fa solo un principio. Ho sentito parlare di nuovi santi e di icone che potremo pregare. Quando un Parlamento considera

l'ordine del giorno, come possiamo leggere, vorrebbe impegnare il Governo ad una necessaria operazione per facilitare la trasparenza in relazione ai bilanci delle fondazioni, degli intermediari finanziari e assicurativi e delle società quotate. Invito il Governo e il relatore

differentemente invece dai primi sette articoli del provvedimento, che hanno visto il nostro voto favorevole. Riteniamo che il falso in bilancio, che pure era stato un argomento di grande discussione, anche nel corso della campagna elettorale, e il solenne impegno della coalizione di centrosinistra laddove avesse vinto le elezioni (anche per chiudere una fase, a nostro avviso, molto negativa della storia di questo Paese), viene invece presentato in questo disegno di legge, o, meglio, viene stravolto stravolto rispetto al testo originario. Sostanzialmente ci appare un compromesso al ribasso che - a nostro avviso - non soddisfa le esigenze che invece c'erano e che, per l'appunto, non sarà positivo rispetto a quello che sarebbe servito. Già nel corso della discussione generale, immaginando, purtroppo, che gli emendamenti che avevamo presentato insieme ad altre forze politiche sarebbero stati respinti, avevo parlato di occasione perduta. Consideriamo sbagliato l'utilizzo del termine «consapevolmente» perché - a nostro avviso - restringe troppo l'area di applicazione della norma. Avevamo anche presentato una serie di emendamenti per sostituire con un termine più ampio la definizione di fatti materiali, riprendendo proprio la dizione del suo testo (la parola «informazioni» ci sembrava più adeguata). un'altra cosa, peraltro in un Parlamento in cui si aumentano le pene su tutto e anzi, in qualche caso, francamente - su questo ha davvero qualche ragione il senatore Manconi - in

una ben altra impostazione da questo Governo e da questa maggioranza parlamentare. il Gruppo di Forza Italia voterà contro questo articolo. Avevamo dato un contributo non irrilevante perché questo articolo divenisse formalmente costituzionale. Vedremo, da qui a qualche anno, se abbiamo torto noi o se avete ragione voi: l'articolo così come scritto - a nostro

che si voglia fare la lotta alla corruzione approvando regole equivoche e non garantendo quegli imprenditori

e, allo stesso tempo, creare un tale allarme, successivamente all'applicazione di queste norme, da distruggere quel minimo residuo di capacità delle piccole e medie imprese.

Io mi auguro che il presidente Renzi voglia veramente portare questo Paese alle elezioni nel 2018. Avremmo così la possibilità nel 2017 di verificare in concreto se questa normativa ha avuto o no una qualsiasi possibilità di seria applicazione nel combattere la corruzione. Io credo di no.

si risponde con il silenzio. Probabilmente non si hanno argomenti da contrapporre; probabilmente quello che diciamo dal punto di vista tecnico coglie nel segno e, nonostante la consapevolezza, gli ordini di scuderia prevalgono. *(Applausi

Signor Presidente, questo emendamento, come il successivo 9.315, tende a introdurre qualche elemento di mitigazione nell'azione di sanzionamento verso le piccole imprese. È evidente che i fatti delittuosi attribuibili al comportamento all'interno delle imprese hanno certamente, dal punto di vista del principio, la stessa valenza; ma dal punto di vista della sostanza, hanno valenze molto differenziate. Si chiede pertanto l'introduzione dell'azione a querela per quanto riguarda le società minori quando sono tutelate con la querela di parte, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale, non si vede perché si debba introdurre l'azione d'ufficio in quanto i principali interessi sono tutelati attraverso la querela di parte.

alle buone pratiche contabili - espressione che nelle relazioni di bilancio viene richiamata ripetutamente - è un elemento di tutela degli interessi dell'impresa, oltre che di buona giustizia.

con il quale in qualche modo si cerca di porre rimedio a quelli che possono essere danni irreversibili nei confronti di piccoli imprenditori e di piccole società.

mi pare che sia un'attività corretta. Mi stupisco dunque che il senatore Buemi, che aveva fatto un buon emendamento, lo ritiri, per cui lo faccio mio e chiedo che venga votato.

di questa maggioranza il senatore Buemi si deve rendere conto che ovviamente la strada del riformismo e del socialismo è definitivamente perduta, perché

Presidente, i prossimi tre emendamenti su cui abbiamo chiesto il voto segreto, tendono a rendere costituzionalmente legittimo il testo del

Presidente, so benissimo che non possiamo più porre rimedio al fatto che si sta tornando agli anni '90, quando i pubblici ministeri - lo sa meglio di me

evitare ciò che la Corte costituzionale vi ha già detto. Anche la collega Ricchiuti ha svolto diversi interventi in merito ai quali fate orecchie da mercante, semplicemente per rispettare un ordine di scuderia.

vi abbiamo offerto la possibilità di rendere tutto legittimo. È un reato tale da poter colpire effettivamente chi compie falso in bilancio

può darsi che non siano applicabili o non possano essere accettate perché facevano parte della riforma del Governo Berlusconi.

Che cosa è avvenuto poi? Per il giustizialismo di alcune fette del Partito Democratico è stato necessario indire una riunione notturna e dai giornali abbiamo appreso la mattina che era stato predisposto un nuovo testo che correggeva quello che il Governo, dopo mesi e anni di studi dei tecnici degli uffici legislativi aveva correttamente fatto.

Vi rendete conto dell'assurdo e dell'irresponsabilità di arrivare, a distanza di qualche mese, a cambiare le carte in tavola senza preoccuparsi degli effetti sull'economia, sulle aziende? Questo è di una scorrettezza unica.

soglie di non punibilità. Se può avere un fondamento di ragionevolezza parlare della tutela delle imprese per evitare che si possa rispondere di un reato anche nei casi in cui non c'è un'alterazione sensibile alla rappresentazione della situazione economica, la reintroduzione di una soglia di non punibilità, come prevista nell'emendamento 9.316, farebbe ripiombare questo Paese nella situazione in cui è da tredici anni, cioè da quando si sono avuti i risultati concreti della legge Berlusconi, cui il senatore Caliendo faceva riferimento, e che - come sappiamo bene tutti

l'amministratore unico, il contabile disonesto sapevano bene che potevano operare più falsi in bilancio, ciascuno dei quali inferiori alla singola soglia di non punibilità, per garantirsi l'impunibilità e i fiumi di denaro che da parte delle società non quotate

coprono ampiamente ogni ragionevole preoccupazione esposta dal senatore Caliendo. Mai più soglie di non punibilità!

il voto favorevole del Movimento 5 Stelle su questo emendamento attiene ad una circostanza che probabilmente può essere condivisa da tutti i colleghi: l'esclusione del riferimento all'Unione europea in relazione ai mercati regolamentati per i quali le società quotate possono essere punibili in caso di falso in bilancio. In sostanza non capiamo perché, nel testo che viene proposto all'esame si faccia riferimento solo ai mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea. Non capiamo perché se, ad esempio, una società quotata, che piazza titoli o altri prodotti finanziari nella Borsa di Hong Kong o di qualsiasi altro Paese al di fuori dell'Unione europea debba avere questa via di fuga, che troviamo francamente poco ragionevole. L'emendamento soppressivo

Grazie, corretta osservanza delle regole, va segnalato anche questo sistema intimidatorio che quel senatore usa costantemente facendo, in maniera non consentita dalle nostre regole, riprese delle votazioni d'Aula, che spingono in termini di sfida a rifiutare questa prevaricazione. È giusto quindi che ognuno voti regolarmente, ma è altrettanto giusto che si smetta di fare queste riprese da parte del senatore Ciampolillo. Le regole valgono per tutti.

Signor Presidente, una volta per tutte, siccome stiamo parlando di anticorruzione e credo che la legalità in quest'Aula non possa assolutamente essere messa in discussione, chiedo chiedo che lei acquisisca immediatamente i video per verificare se nella votazione dell'emendamento 10.311, che è passato per soli tre voti, è stato inserito anche quel voto. Le chiedo quindi gentilmente di annullare la votazione e di ripeterla, perché non può essere messa in nessun momento in discussione la legalità all'interno di questa istituzione. Lei è il garante della legalità in questo momento, quindi le chiedo gentilmente, dopo aver ritirato tutte le tessere dei senatori che non sono presenti, di ripetere la votazione in questione, onde fugare qualsiasi altro dubbio.

i video anch'io, perché non è possibile e non è accettabile che venga svilita la legalità all'interno dell'Aula del Senato della Repubblica. È inaccettabile per tutti. Anche per voi.

profili che secondo me sono inaccettabili, soprattutto oggi che stiamo votando questo disegno di legge. Vorrei chiederle una sua opinione, signor rispetto al fatto che un senatore della Repubblica italiana indirizzi ai nostri banchi epiteti come «imbecille», «buffone» e frasi come «non saresti eletto neanche nel condominio di casa tua». Questo, secondo me, è gravissimo e il senatore Aracri dovrebbe essere allontanato come siamo stati cacciati noi da questa Aula

i senatori del PD ci hanno suggerito di non protestare contro il voto truffaldino del senatore Aracri perché quel voto avrebbe favorito la nostra votazione. Noi a questo non ci stiamo.

che possono notare quanto sia scoppiettante la dialettica parlamentare.

Presidente, l'ostruzionismo è una pratica ammessa in quest'Aula e io, quando alcune forze politiche attuano

uno del senatore Aracri, che avrebbe votato per il senatore Tarquinio, e l'altro del senatore Ciampolillo, che continua, da quand'è venuto in questa Aula, a riprendere con foto. *(Commenti Sono due inadempimenti altrettanto censurabili e credo che, detto questo a lei e affidata la questione alla sua sensibilità

che prevede il reato di corruzione, mentre nella sostanza il Movimento 5 Stelle questa mattina si è dato ad una pratica di ostruzionismo miserevole che non si conviene alla loro forza politica.

senatori Segretari abbiamo ritirato la tessera del senatore Tarquinio,

«In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente,» - quindi lei - «apprezzate le circostanze,» - che sono evidenti - «può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico». Grazie, signor Presidente.

avallare questo comportamento? Noi stiamo segnalando delle irregolarità. Il Consiglio di Presidenza continua a non dichiarare alcun tipo di pronunciamento su tali

auspicabilmente, con lo stesso garbo, forse potrebbe accogliere la richiesta del Gruppo. Vede con quanta leggerezza glielo chiedo? I miei colleghi sono stati più irruenti. *(Commenti del senatore

ogni minimo dubbio. Se è facile dissiparlo, perché non farlo? Vede con quanta leggerezza glielo chiedo? Spero che voglia accogliere questa leggerezza con altrettanta tranquillità. Con altrettanta leggerezza, le rispondo che, come lei può ben verificare, il voto di differenza non è assolutamente influente rispetto alla votazione. SANTANGELO *(M5S)*.

permettere, qualora l'autorità giudiziaria lo ritenga opportuno nell'ambito delle indagini, di disporre intercettazioni telefoniche senza mettere mano alla pena massima. Proponiamo dunque la modifica del codice di procedura penale per fare in modo che in tutti i casi in cui sia necessario, senza aver messo mano alla pena massima, sia possibile disporre intercettazioni telefoniche. Sappiamo bene che probabilmente questo tipo di strumento investigativo nel caso di specie

all'autorità giudiziaria la possibilità di utilizzare lo strumento delle intercettazioni ambientali e telefoniche anche nel caso di falso in bilancio e senza mettere mano alla pena edittale. Credo sia

apprezzo senz'altro il suo intento di recepire in un emendamento i criteri formulati dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione nella lettera indirizzata il 28 gennaio scorso ai Presidenti delle Camere.

stiamo parlando di quegli strumenti che nella lotta alla corruzione tutti quanti sappiamo essere necessari, cioè delle iniziative legislative che, al di là dell'aumento delle pene, possono dare alle autorità inquirenti strumenti efficaci per la scoperta e la lotta effettiva al fenomeno corruttivo. Si tratta di proposte, dal nostro punto di vista, tra le più fondanti che questo Parlamento avrebbe l'occasione di esaminare. Mi riferisco alla possibilità di utilizzare, in fase di investigativa ed in maniera coordinata con l'autorità giudiziaria, e quindi non a strascico e alla mercé delle singole iniziative della polizia giudiziaria, le figure, già

del giorno, omesso l'*incipit*, prevede che il Senato: «Premesso: che la repressione dei fatti di corruzione deve costituire una priorità di azione di questa legislatura, come peraltro è stato più volte dichiarato dal Governo; che il potenziamento degli strumenti di indagine è passaggio necessario al recupero di una maggiore effettività del sistema penale su questo versante criminale; che nel contrasto di altre forme di criminalità, non più gravi in termini di costi sociali, è stata positivamente sperimentata l'efficacia delle cosiddette operazioni sotto copertura, da parte di agenti di polizia giudiziaria, per giungere all'accertamento di episodi corruttivi che, altrimenti, resterebbero impuniti raccomanda al Governo di valutare l'estensione delle previsioni dell'articolo 9

314, 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale, commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Sono costretto ad intervenire perché non abbiamo una pubblica amministrazione marcia. Signor Vice Ministro, se così fosse, la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha la responsabilità dell'intero sistema della pubblica amministrazione, probabilmente è consapevole di fatti che a noi sfuggono.

di corruzione! Lei sa meglio di me quanti processi ci sono stati in questo Paese, ma non negli ultimi dieci anni: negli ultimi quarant'anni, da quando c'è la Repubblica, addirittura dal 1946. Mi volete dire quando ci sono stati questi enormi casi di corruzione nella pubblica amministrazione? *(Commenti del

Sapete benissimo che alcuni senatori sono convocati dalla procura della Repubblica di Roma a causa vostra. Io vi difendo, e ritengo illegittimi quegli avvisi a persone informate dei fatti inviati ai senatori.

ciascuno! Se nella pubblica amministrazione - parlo con dati di fatto, certificati - non ci sono episodi di corruzione generalizzata tali da giustificare l'agente provocatore, siete falsi. Portate un elemento a sostegno della vostra tesi! E mi meraviglia che il Partito Democratico, che esprime il Presidente del Consiglio, possa accettare una cosa del genere.

difendete quella che è l'organizzazione del nostro Paese, dello Stato del nostro Paese! Come fate ad accettare un'ipotesi del genere, solo per garantirvi qualche voto nei voti segreti? Ma è assurdo!

Immagino imprese, politici o altri che arrivano con la tangente e non sanno se fidarsi o meno. Vorrei però sottolineare una cosa che ha detto il senatore Caliendo e che secondo me è molto grave,

perché dei senatori della Repubblica vengono convocati dalla procura e per riferire in merito a che cosa, visto che riguarda, come ha detto il senatore Caliendo, se è vero quello che ha affermato... Senatore Caliendo, le sto chiedendo, siccome lei ha affermato una cosa, che, se è vera... Io immagino che sia vera. Lei riferisce che dei senatori sono stati convocati dalla procura della Repubblica per colpa del nostro Gruppo; così ci è stato detto e lei l'ha detto qui pubblicamente in quest'Aula. Chiediamo allora che pubblicamente in quest'Aula si spieghi qual è il motivo di questa convocazione.

Sento parlare di un ordine del giorno in cui si farebbe riferimento all'agente provocatore. Io avrei piacere di leggerlo, signor Presidente, sì da poter intervenire, se del caso, con una conoscenza del contenuto dell'ordine del giorno stesso. In più di un'occasione la Presidenza ha chiesto, su cose molto più semplici e meno corpose di un ordine del giorno, che si desse la possibilità ai senatori di leggere. Io gradirei che la Presidenza volesse usare questa cortesia anche in questo caso, perché una cosa è il cosiddetto agente sotto copertura, cosa completamente diversa è l'agente provocatore, in ordine al quale credo, signor Presidente, che anche ella ricorderà i fiumi di giurisprudenza e di dottrina che vi sono in ordine alla non praticabilità di questa figura nel nostro ordinamento giuridico. Quindi la pregherei di consentire ai senatori di leggere questo ordine del giorno, riservandomi evidentemente di richiedere la parola per intervenire. una seconda cosa, che riguarda la questione che è stata sollevata dal senatore Caliendo e ripresa dal senatore Crimi.

Immagino che si ravvisi lì un attentato agli organi costituzionali, che si sostanzierebbe nell'avere impedito, in tutto o in parte, il corretto funzionamento di detti organi. In ragione di questa ipotesi di reato la procura della Repubblica starebbe svolgendo delle indagini, assumendo a sommarie informazioni i senatori. Io non so se questo sia vero e no ma, signor Presidente, ella dovrebbe assumere le corrette iniziative al fine di verificare se ciò stia realmente accadendo e se, nell'ambito della legittima azione della magistratura, sia ravvisabile un atteggiamento invasivo rispetto all'autonomia del Senato. È evidente, signor Presidente, che tutto ciò non avrebbe senso nel caso in cui la denuncia alla procura della Repubblica Repubblica trovasse nella Presidenza, cioè in lei, la sua origine. È chiaro, infatti, che in quel caso ella, come Presidente del Senato, avrebbe assolto all'obbligo di denuncia, doveroso per la sua qualità, e avrebbe investito del fatto la procura della Repubblica.

il problema aprirebbe degli scenari sotto certi profili inquietanti.

e non rientrando nella responsabilità di chi ha l'obbligo di denunciare la valutazione in ordine ai dettagli del fatto, essendo l'obbligato alla denuncia semplicemente tenuto a valutare il fatto e a investire l'organo competente, questo avrebbe dei risvolti, ahimè non positivi, per la Presidenza del Senato e, per converso, per l'intero Senato. Così come poco fa si sono svolte una serie di proteste dagli appartenenti al Movimento 5 Stelle. Una riguardava un voto che si asseriva essere stato dato da un senatore per conto di un altro. Si è fatto un ragionamento sulla legalità. Immagino che, nel fare questo ragionamento sulla legalità, si sia immaginata una non regolarità della votazione e conseguentemente, forse, anche una una ipotesi di falsità in ordine all'espressione del voto. Io so bene che ella ha applicato a questa votazione la cosiddetta prova di resistenza. In altri termini, essendosi quella votazione risolta per tre voti di distacco, il voto eventualmente annullabile non influiva sull'esito della votazione. Ciò riguarda la regolarità della votazione, ma non l'atto espressivo del voto. Sostanzialmente, in attesa di poter leggere l'ordine del giorno

quanto sta realmente accadendo alla procura della Repubblica di Roma: se, effettivamente, sia in atto un procedimento in ordine a un fatto rispetto alla cui esistenza nessuno può far finta di niente. In ordine a quel fatto, infatti, diversi esponenti del Movimento 5 Stelle sono stati sanzionati dal Consiglio di Presidenza, il che equivale a dire che il Consiglio di Presidenza era perfettamente a conoscenza, nel suo complesso, di quello che era accaduto, con quanto inevitabilmente ne dovesse conseguire nel caso in cui non si dovesse far rispettare l'autonomia del Senato e la corretta valutazione di atteggiamenti politici esasperati, sbagliati ed illegittimi, se si vuole, ma che in linea di massima, come diceva prima il senatore Caliendo, pur vibratamente contestato dal Movimento 5 Stelle, mi pare siano connotati esclusivamente dalla politica.

comunque che sia importante parlare di questa vicenda estremamente delicata, che è già stata affrontata non soltanto durante l'esame in Commissione, ma in anni di approfondimenti giurisprudenziali ed anche dottrinari. Si tratta delle operazioni sotto copertura,

si tratta di istituti molto diversi, che destano giustamente delle perplessità. Peraltro voglio ricordare che, per quanto concerne le operazioni sotto copertura, già esiste una normativa italiana specifica in materia, quantomeno dal 2006 (la legge n. 246 del 2006), che fa espressamente riferimento a queste operazioni sotto copertura

estendere questo istituto dell'operazione sotto copertura anche alla materia dei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare della concussione e della corruzione. così com'era impostato, quell'emendamento 1.0.304, in particolare al primo comma, qualche perplessità me l'ha destata anche ora, così come già in sede di Commissione, proprio per la configurazione tecnica e giuridica, perché interviene su una materia diversa, che ha anche delle prospettazioni di comportamenti diversi, che male si adatterebbero alla fattispecie della corruzione e della concussione in particolare. Quando infatti si fa riferimento, nella legge n. 246 del 2006, alla possibilità di dare rifugio e prestare assistenza agli associati per reati che concernono armi, munizioni ed esplosivi, faccio fatica a dare un'interpretazione lineare e corretta di questo inserimento.

fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti» di corruzione e concussione, a comportamenti che si limitano alla simulazione di accordarsi o alla partecipazione materiale alla commissione, cosa ben diversa dall'istituto giuridico dell'agente provocatore, peraltro ampiamente utilizzato da molto tempo negli Stati di diritto anglosassone, che nel nostro ordinamento creerebbe problemi consistenti non soltanto per l'aspetto normativo-giuridico, ma anche per gli aspetti elencati di fatto dal senatore Caliendo. concludo dicendo che, per quanto riguarda la figura dell'agente provocatore, se in sede di emendamento 1.0.302 voterò contro per la pericolosità in sé di questa norma, per com'è impostata, di fronte all'ordine del giorno, come quello preannunciato, che fa riferimento al secondo comma dell'emendamento 1.0.304, credo che si possa consentire a dare un parere e un voto favorevole proprio perché si inserisce nell'ordinamento, adeguando alla fattispecie e proponendo al Governo di adeguare questi comportamenti di tutela della pubblica amministrazione dai delitti di corruzione e concussione, così come è stato fatto già per i delitti di mafia e terrorismo.

Signor Presidente, l'ordine del giorno è una raccomandazione a valutare.

L'argomento è quello delle operazioni sotto copertura, non quello dell'agente provocatore. Mi pare che questa sia una differenza essenziale che in alcuni interventi non è stata evidenziata.

accade un episodio che dimostra come spesso vi sia confusione nella gestione dei lavori d'Aula. Si è data lettura di un ordine del giorno. Sulla base di questa lettura, in un'Aula che possiamo definire «parlante», non tutti i passaggi dell'ordine del giorno sono stati percepiti. Dopodiché, senza che i senatori avessero la possibilità di leggere l'ordine del giorno, lo si è messo in votazione affermando che vi era il parere favorevole del relatore e del Governo. Correggo: non si è messo in votazione. Si è soltanto acquisito il parere.

ha portato il senatore Caliendo a un intervento molto appassionato, che io condivido dall'inizio fino alla fine, sul presupposto che si stesse cercando di introdurre nel nostro ordinamento la figura dell'agente provocatore. Letto l'ordine del giorno, che sostanzialmente richiede un'estensione anche alla materia della corruzione dei cosiddetti agenti sotto copertura, la richiesta viene accolta dal Governo come raccomandazione a valutarne l'opportunità. Il Gruppo di Forza Italia non esprime contrarietà, ribadendo però un concetto di fondo. L'agente sotto copertura è previsto nel nostro ordinamento con riferimento ai reati di tipo associativo o a quelli che normalmente fanno richiamo e si correlano ad una possibile forma associativa. È chiaro che lo

di quello che accade per i reati contro la pubblica amministrazione, in cui se per un verso è vero che vi sono dei sistemi corruttivi (penso alle grandi opere, per cui questa norma avrebbe un senso),

dal telefono, nel valutare l'opportunità e l'esito di questa raccomandazione, tenga presente, non solo quanto ho fin qui esposto in ordine ai reati associativi, associativi, ma anche questo: in reati per lo più sinallagmatici l'agente sotto copertura corre il rischio di diventare un agente provocatore. Conseguentemente, mi auguro che questo elemento di fortissimo rischio, che snaturerebbe la figura dell'agente sotto copertura, nella sostanza in un agente provocatore, con un danno enorme per il nostro ordinamento, possa essere sottoposta possa essere sottoposta alla particolare attenzione del Governo nel valutare le iniziative che riterrà di voler far adottare.

Presidente, è simile, ma manca, rispetto a quello trasformato in ordine del giorno, un comma che dà ulteriori specificazioni. Questo è un emendamento che, prendendo atto dell'accoglimento dell'ordine del giorno del Governo sulla materia, seppur nell'ipotesi della valutazione dell'opportunità dell'opportunità di introdurre la figura dell'agente sotto copertura, riteniamo opportuno mettere al voto, anche come gesto di testimonianza. Ci tengo a specificare quello che sembra essere stato chiarito, cioè questo fraintendimento tra la figura

all'intendimento che il Governo sembra aver accolto.

o eventualmente intervenire su questo tema, devo avere la possibilità di aprire il codice - che qui peraltro non viene dato in dotazione - e andare a cercarlo, per vedere a quale norma del codice penale non menzionata

ma, ancorché riconosca a lei tutta l'autorevolezza della sua funzione, mi permetterei sommessamente di non consentirle di mettere in discussione la mia attività

che può venire da parte di chi, come anche noi, tiene alla tutela dei diritti e dei principi costituzionali, dal diritto alla *privacy* a tutto quello che vogliamo mettere sul piatto. Quindi, questo istituto di primo acchito può sembrare certamente eccessivamente incisivo. e vi chiedo: non è forse arrivato il momento che questo Paese adotti strumenti di tipo investigativo - attenzione, siamo nell'ambito investigativo

da parte della classe dirigente della politica partitica, non è forse il momento di provare? Almeno facciamolo per un periodo di tempo: ripuliamo la pubblica amministrazione a tutti i livelli

e su delega della procura. Non stiamo lasciando il campo libero ad una pesca a strascico, che certamente potrebbe avere effetti paradossalmente contrari. Non vogliamo instillare il panico, se un certo tipo di panico per le persone disoneste avremmo tutto il piacere di diffonderlo, sulla base dell'idea che se in tutti gli uffici della pubblica amministrazione italiana

se voleste adottare questo istituto. Perché non volete farlo, allora? Per il timore nascosto dalla valutazione ipocrita che così bloccheremmo la pubblica amministrazione. Già so che ascolteremo questo tipo di interventi e osservazioni critiche: così congeleremmo gli amministratori e i dirigenti perché avrebbero

deve arrivare, perché altrimenti non ne usciamo - il tempo dell'onestà, e siccome abbiamo detto tutti che l'aumento delle pene magari non è sufficiente, usiamo questi strumenti che sono efficaci. usiamo questi strumenti che sono efficaci. Facciamo in modo che chi è in situazioni di potere e di gestione del denaro pubblico abbia il sacrosanto timore non solo della pena, che può essere la più severa possibile, ma di non sapere come muoversi. Mettiamolo nell'imbarazzo di non cedere alla tentazione. Facciamo qualcosa di utile anche per gli amministratori onesti, perché chi svolge il suo ruolo adeguatamente e con senso civico e responsabile non credo abbia nulla da temere. Questa è un'occasione storica; è una proposta che noi ci aspettiamo possa non essere accolta oggi, anche se insistiamo sulla grande occasione che il Senato potrebbe avere nell'introduzione di questo istituto. di questo istituto. Colleghi, vi invito a leggere il testo dell'emendamento. La finalità dell'intervento dell'agente provocatore è quella di cogliere gli autori in flagranza o comunque di farli punire. Sono identificati i reati per i quali sarebbe opportuno autorizzare la procura a introdurre

disciplinari da parte del Consiglio di Presidenza del Senato, mentre chi dall'inizio della legislatura continua a violare la prima regola, quella che dovrebbe permettere di guardare negli occhi i cittadini uscendo da quest'Aula, questo, Presidente, ma capisce bene che è qualcosa di insopportabile agli occhi dei vostri elettori, non solo dei nostri. Non ci interessano però gli elettori. Non ne possiamo più. Il Movimento 5 Stelle ancora una volta vi offre un'occasione su un piatto d'argento. Approfittatene; approfittiamone. Le uniche osservazioni che potranno essere fatte saranno quelle alle quali ho cercato in maniera anticipata di replicare: si potrà dire che non ci sono corpi speciali per l'anticorruzione. Mentre oggi per i reati contro il terrorismo, la mafia, la pedopornografia ci sono reparti specializzati, per

una premessa. Il senatore Buccarella ha fatto riferimento ad una votazione che sarebbe stata fatta precedentemente per conto terzi come un dato di illegalità.

Il senatore Buccarella dice che deve arrivare il tempo dell'onestà, ma l'onestà è un valore che in uno Stato si valuta con la legalità. Quando si fanno delle leggi l'onestà pare coincidere con la legalità. Il problema, quindi, non è fare un riferimento suggestivo ma propagandistico all'onestà, ma stabilire se quello che si propone è in linea con il nostro ordinamento, sia costituzionale che settoriale.

deve indurre o istigare un pubblico ufficiale alla commissione di un reato, cosa conta che quel pubblico ufficiale sia già indagato, vale a dire abbia già commesso un reato? E che rileva l'agente provocatore in ordine al reato già commesso?

perché la giurisprudenza, che il senatore Buccarella ben dovrebbe conoscere, si è sempre palesata contro l'agente provocatore?

di commissione o sta per essere commesso, ma è una persona che induce o istiga altro soggetto a commettere un reato. Il pubblico ufficiale vive per i fatti suoi, viene avvicinato dall'agente provocatore che, in cambio di qualcosa, gli offre una somma di denaro. Il pubblico ufficiale cade in tentazione e da lì, all'interno di una grande finzione, risponde di un reato mentre l'istigatore non risponde di nulla.

nel caso di raggiungimento dell'accordo, vi è il concorso nel reato; mentre, nel caso di non raggiungimento dell'accordo per un determinato tipo di reati, vi è la misura di sicurezza. E quindi, il nostro ordinamento settoriale è assolutamente contrario all'agente provocatore. Certo, c'è il dato pratico. L'agente provocatore sarebbe in grado di accelerare le indagini rispetto ad un fenomeno grave come la corruzione. ha la facoltà di non rispondere all'interrogatorio e, ove dovesse rispondere, può mentire, salvo il limite della calunnia. Potremmo, per ipotesi, modificare anche queste norme e stabilire l'obbligo di rispondere e di dire il vero. Che importa poi se l'articolo 24 della Costituzione garantisce all'imputato il diritto al silenzio? In questo modo le indagini su un determinato reato. Il risultato pratico sarebbe così importante da consentirci una scrollata di spalle rispetto ad una violazione ordinamentale, e ancora. Nessuno può sottoporre l'imputato ad un esame psicologico. Forse l'unico esame psicologico previsto nel nostro codice è quello dell'interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria e ripeto forse, Il nostro ordinamento vieta, ad oggi, le lesioni, la violenza privata e quant'altro, anche finalizzate ad estorcere una confessione.

Ma pensate cosa accadrebbe se introducessimo la tortura nel nostro ordinamento. Faremmo prima, faremmo più in fretta, la gente parlerebbe e noi riusciremmo ad acquisire prove. Perché sto facendo questo discorso e ne potrei fare tanti e tanti altri ancora? Perché nel nostro ordinamento legalità significa rispetto delle regole generali e delle regole costituzionali. Infatti - cosa che forse il senatore Buccarella, nell'enfasi del suo discorso politico, ha dimenticato il codice di procedura penale veniva definito da Carnelutti come il codice di garanzia, cioè come il codice posto a tutela delle ragioni del più debole, cioè dell'imputato, e che sul piano del rispetto delle garanzie, coperte tutte dalla nostra Carta costituzionale, non sono ammesse scorciatoie; non è consentito a nessuno, per raggiungere un risultato, di violare il nostro ordinamento. Tutto ciò che voi state dicendo può andare bene per una propaganda, invero rozza, ma non va bene in queste Aule dove, essendo voi legislatori, almeno i principi generali del diritto dovreste conoscere. Accontentatevi della raccomandazione accolta dal Governo. Accontentatevi dell'agente sotto copertura. Prendete atto dei limiti che la nostra Costituzione e il nostro ordinamento vi pongono. Lasciate la strada della propaganda. A molti di voi che sono molto più giovani - ahimè - di me, vorrei ricordare che, quando c'era il fenomeno del terrorismo, non sono state prese scorciatoie e non sono state fatte leggi speciali.

ma sul piano delle garanzie individuali nulla venne toccato. Quella legge sarebbe un cucchiaino di miele - per così dire - rispetto a quanto voi state legiferando in questi tempi. Siete così presi dalla voglia di portare demagogici risultati alla popolazione che vi dimenticate dei principi generali del nostro ordinamento. È per questo, signor Presidente, che il Gruppo di Forza Italia voterà contro questo emendamento: pur potendo comprendere

senatore D'Ambrosio Lettieri)*. E, quando busserà a casa loro, si renderanno conto del valore di tutte le battaglie garantiste che voi, per motivi molto chiari, avete contrastato in questi anni e che erano il vostro bagaglio,

Provocatoriamente chiedo: come potrebbe essere affrontato il problema legato ad un pubblico ufficiale che momentaneamente accondiscende al tentativo, da parte dell'agente provocatore, e poi successivamente denuncia il comportamento del soggetto provocante alla procura della Repubblica? In base al nostro ordinamento, quale sarebbe il

riferisco alla dichiarata non procedibilità o improponibilità del mio emendamento che ha affrontato il tema dell'informatore interno, ossia del pubblico ufficiale presente in un ufficio nel quale si si svolge un'attività che si presume criminosa, il quale sente il dovere civico di segnalare all'attività giudiziaria il comportamento da lui ritenuto non conforme alle regole.

poi sottolineare la differenza notevole che esiste fra i due istituti giuridici e ricordare come questo strumento è certamente in uso da diverso tempo nei sistemi di diritto anglosassone, dove non sempre ha dato un'ottima prova di sé. sono stati dei casi certamente positivi, ma anche altri pericolosi e casi di ricatti, di estorsioni e concussioni nel nostro ordinamento, che hanno fatto discutere dottrina e giurisprudenza.

assolutamente insufficiente e non consenta di dire che si introduce un istituto giuridico nuovo così rilevante e pregnante, che va così a fondo relativamente alla libertà delle persone e al corretto rapporto processuale. Ci sarebbe la necessità forte di reimpostarlo e di prevedere delle norme attorno ad esso molto particolari, che hanno a che fare non soltanto con l'impostazione secca della promessa o dell'offerta di denaro.

dell'esigenza di avere una capacità, un *team* o una *task force* di*intelligence* in questa materia si fosse fatta carico addirittura la Convenzione ONU anticorruzione, che proponeva agli Stati firmatari

Governo Berlusconi. In sostanza, vorrei dire che, se comprendo la necessità di pensare ad un agente provocatore, faccio però fatica a votare un emendamento di questo tipo, proprio da un punto di vista tecnico, sostanziale e processuale. Ora, se dovesse essere proposto al Governo di valutare, assieme alla figura dell'operazione sotto copertura, anche la figura dell'agente provocatore, per la complessità reale della materia, soprattutto dal punto di vista costituzionale e processuale, potrebbe essere fatto un passo in avanti e non ci sarebbero spaccature o valutazioni ipocrite, com'è stato detto. Se ci fosse questo passaggio, potrebbe essere positivo. In caso contrario, su questo tema, così come impostato e risolto dal primo comma dell'emendamento 1.0.302, credo che non si potrà votare a favore.

potrebbe rendere efficace tutto il provvedimento che è attenzionato dal Senato in questo momento, per cui ne sottolineo l'importanza. mi trattengo ancora pochi secondi per ricordare che su questo provvedimento, cioè sul DASPO per corrotti e corruttori, è stata fatta una promessa a 60 milioni di cittadini non dal Movimento 5 Stelle, ma dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. Spesso si è detto che l'aumento delle pene non si trasforma in un aumento di efficacia della portata di deterrenza della norma. Per un certo verso sono anche d'accordo. Secondo me, è necessario, ma non è sufficiente. Ecco, qui parliamo non di aumento delle pene, delle pene, ma di una pena accessoria, che può essere ancora più efficace della sanzione detentiva. Per questo siamo convinti che l'introduzione di una norma di questo tipo avrebbe una straordinaria rilevanza dal punto di vista dell'effetto di deterrenza nei confronti del reato di corruzione nel nostro Paese. Detto questo, chiedo chiedo al Governo e al relatore se intendano considerare una possibilità di riformulazione della seconda parte dell'emendamento, per